*dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*: "Conversione in legge del decreto‑legge 5 febbraio 2009, n. 4, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario"

link apre una nuova finestra"). Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato modifiche ed integrazioni al calendario della settimana corrente. All'ordine del giorno della seduta odierna è stato posto il disegno di legge n. 1369, recante "Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione". Il termine per la presentazione degli emendamenti, già comunicato ai Gruppi e ormai decorso, è stato fissato per le ore 18. I tempi per la discussione del provvedimento sono stati ripartiti, per complessive cinque ore, nel modo seguente, al fine di concludere le votazioni entro questa notte, presumibilmente intorno alle 24 o anche oltre, se necessario.

Ai dissenzienti sono attribuiti complessivamente 10 minuti. Il voto finale sull'articolo unico del disegno di legge avrà pertanto luogo immediatamente a conclusione delle dichiarazioni di voto.

Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, questo provvedimento, che reca una normativa tendente a fissare un principio fino all'approvazione di una legge organica, non è consentito in alcun modo sospendere l'idratazione e l'alimentazione, non ha potuto compiere il cammino conclusivo nella Commissione in sede referente. Abbiamo avuto, nei tempi concessi, la presentazione di quattro pregiudiziali e di quattro sospensive, per cui è stato possibile solo procedere ad alcuni interventi in discussione generale, che hanno consentito quantomeno un forte approfondimento e una diversificazione di due posizioni su questo argomento. Ricordo, com'è stato ricordato in quella sede, il nucleo cruciale della legge su questo argomento riguarda proprio questo elemento, e quindi riteniamo che l'approfondita discussione e il confronto in Aula - com'è stato richiesto - valgano a giungere a delle decisioni conclusive. Grazie, signor Presidente. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Tomassini, non essendo stato concluso l'esame in Commissione, il disegno di legge n. 1369 sarà discusso nel testo del proponente senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento. Comunico che sono state presentate questioni pregiudiziali e sospensive. Ha facoltà di parlare la senatrice Bonino per illustrare la questione pregiudiziale QP1.

quando un Governo è capace di inventare falsità a reti unificate, trasformarle in decreto e poi portarle per essere timbrate in un Parlamento addomesticato e ricattato dal pietismo televisivo,

BONINO *(PD)*. Uno Stato che entra nel letto dei pazienti, ovviamente a fin di bene (che è sempre stata la giustificazione di tutti gli orrori della storia e il fondamento di ogni totalitarismo), e che tende a non uscirne più, se qualcuno non lo ferma: tutto questo dovrebbe terrorizzarci e terrorizzarvi. Solo in Italia, pare, chi pure si proclama liberale può non vederlo. E questo, oltre il calvario di una famiglia, è ciò che in queste ore disperanti è in gioco anche per coloro che dicono di non avere opinioni sulla situazione Englaro e si credono fuori dalla tragedia. Non lo siamo. Non lo siete. Oggi il combinato disposto di un'accelerazione incredibile dei lavori parlamentari e della trasformazione di un decreto-legge in un disegno di legge, in un Parlamento che ritiene che 50 minuti siano sufficienti a togliere la libertà ai cittadini, tutti quanti (è la libertà ai cittadini che è in gioco!),

state dando un ulteriore colpo, durissimo, al già pesantemente distrutto Stato di diritto nel nostro Paese. Per questo la rivoluzione di un padre, accanto al quale noi siamo. E ricordate, signori della maggioranza, che, quando uno dice "io non lo farei" e ciò improvvisamente diventa "e quindi nessuno lo deve fare", questo è lo Stato totalitario, questo è lo Stato etico, questo è l'inizio che voi ci presentate.

Signor Presidente, sono obbligato a leggere dalla brevità inverosimile a cui siamo stati costretti. Il principio fondamentale della distinzione e del reciproco rispetto tra poteri e organi dello Stato non dovrebbe consentire di approvare un provvedimento di legge avente il solo fine precipuo di disattendere la soluzione che sia stata già risolta con decisione giudiziaria definitiva adottata sulla base dei principi, anche costituzionali, desumibili dall'ordinamento giuridico vigente. La Corte di cassazione (sezione I civile, n. 21748 del 2007) ha stabilito che il legale rappresentante che chiede l'interruzione del trattamento vitale ... agire nell'esclusivo interesse dell'incapace; e, nella ricerca del *best interest*, deve decidere non "al posto" dell'incapace né "per" l'incapace, ma "con" l'incapace: quindi, ricostruendo la presunta volontà del paziente incosciente, già adulto prima di cadere in tale stato, tenendo conto dei desideri da lui espressi prima della perdita della coscienza...». Pertanto, l'interruzione del trattamento può venire disposta soltanto: "*a)* quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre che la persona abbia la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e *b)* sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, concordanti e convincenti". Desta gravi perplessità l'adozione di una disciplina dichiaratamente provvisoria e a tempo indeterminato delle modalità di tutela di diritti della persona, costituzionalmente garantiti dal combinato disposto degli articoli 3, 13 e 32 della Costituzione: disciplina altresì circoscritta alle persone che non siano più in grado di manifestare la propria volontà in ordine ad atti costrittivi di disposizione del loro corpo. Peraltro, la mancanza di un termine chiaramente individuabile alla disciplina transitoria, in caso di inerzia del legislatore - inerzia reiteratamente riscontrata nella materia in questione - renderebbe eterna la normativa transitoria. Nel caso in esame, invece, la soluzione transitoria individuata (cioè il divieto di sospensione *tout court*) pone nel nulla lo stesso disegno di legge sul testamento biologico. Si tratta, quindi, di un disegno di legge in sé contraddittorio: quale interesse vi sarebbe infatti a varare una normativa sulle dichiarazioni anticipate in presenza di un divieto così drastico, che le supera e le vanifica? Non solo: il legislatore dice che la disciplina che dovrà entrare in vigore a regime dovrà essere completa e organica, ponendo come vincolo condizioni senza le quali non si verificherebbe la cessazione

qualificata come disciplina della "fine vita" appare assolutamente indeterminato e forse anche difficilmente determinabile, potendosi in estremo dire non suscettibile, per sua natura, di alcuna regolamentazione normativa nella relazione del Governo al disegno di legge n. 1369 si legge che: "con il presente disegno di legge si modifica l'assetto normativo della materia per l'aspetto riguardante chi non è in grado di provvedere a se stesso, senza peraltro incidere su alcun giudicato, in quanto, oltre alla considerazione che rispetto ad un provvedimento di volontaria giurisdizione è inappropriato parlare di giudicato, in ogni caso tale giudicato non può coprire anche situazioni sorte sulla base di una successiva normativa".

Va rilevato, viceversa, che la sentenza della Corte di cassazione rappresenti un chiaro e palese giudicato: la Cassazione ha cioè "definitivamente" riconosciuto un diritto soggettivo assoluto, ascrivibile ai principi degli articoli 13 e 32 della Costituzione.

l'esercizio di un diritto soggettivo, riconosciuto dalla suprema giurisprudenza. Il legislatore mantiene sempre la possibilità ed il dovere - ancorché lo ritenga - di intervenire *pro futuro*. nell' Atto Senato n. 1369 l'idratazione e l'alimentazione vengono - *ope legis* - qualificate sempre e comunque come "forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze". Il disegno di legge non le concepisce altro che in questo modo, pur non essendosi raggiunta, né in altri ordinamenti né dal punto di vista della scienza medica, una chiara e definita opzione verso l'esclusione o l'inclusione delle stesse tra i trattamenti medici. L'atto Senato n. 1369 in esame non opera alcuna distinzione di situazioni difformi, racchiudendole tutte in un medesimo trattamento obbligatorio indifferenziato. Una lettura cieca ed astratta del precetto vieterebbe persino una sospensione temporanea di idratazione ed alimentazione. Vengono imposte sempre idratazione e nutrimento a tutti coloro che non sono in grado di provvedere a se stessi, qualunque sia la valutazione dei medici e dei soggetti circa le terapie da adottare nel singolo caso. Poiché l'impostazione dell'articolo 32 della Costituzione fa riferimento sempre alla persona, appare evidente che dinnanzi ad un trattamento indifferenziato che nega in radice il senso stesso della scienza medica, che valuta le condizioni di ciascun individuo e su quelle calibra le cure, ci troviamo in presenza di un conflitto sia col principio di ragionevolezza che con la lettera stessa della Costituzione. Peraltro, ponendosi dal giorno della pubblicazione della legge approvata un divieto secco ed assoluto di sospensione, nulla venendo detto sulle situazioni di sospensione in essere, è evidente che si toglie qualunque spazio alla scienza medica circa la possibilità di ripristinare, senza danno, ciò che è stato interrotto per un dato periodo di tempo. Nulla si afferma circa le conseguenze che tale ripristino ripristino in forza di legge determinerebbe sulla salute del singolo paziente, potendosi paradossalmente ed astrattamente determinare proprio un danno gravissimo in assenza di valutazione del medico circa la ripresa di determinati trattamenti. Anche in questo caso l'indifferenziata ed irragionevole uniformità del divieto, nonché la compressione dei diritti del paziente

Rientrano, in un concetto tanto sommariamente e sciattamente delineato, anche coloro che, pur non potendo provvedere a se stessi, possono esprimere la propria volontà? Sono interessati dal divieto anche coloro che solo temporaneamente non possono "provvedere a se stessi" o solo coloro che versano in stato vegetativo permanente? L'indeterminatezza, che non costituisce aspetto secondario legge, coinvolge anche, sul lato "attivo", colui che "assiste" tali persone ed al quale è imposto il divieto di procedere a sospensione. Nulla il disegno di legge dice per circoscrivere il soggetto che "assiste": formula così ampia e vaga da finire, ove applicata pedissequamente, con l'incentivare quella stessa pratica eutanasica che pure si dice di voler assolutamente la stessa procedura utilizzata sul piano parlamentare per approvare la disposizione in oggetto, la relazione introduttiva all'Atto Senato n. 1369 ed infine i lavori preparatori della stessa qualificano chiaramente il provvedimento, per un singolo e specifico caso e contro una singola e specifica sentenza/decreto, situazione della quale non può non tenersi conto ai fini della costituzionalità della stessa, per quanto l'ultimo capoverso della relazione assurdamente si avventuri a negarlo. Il soggetto in questione ha visto riconosciuta, nelle forme e secondo le procedure previste dalla legge vigente, il riconoscimento della propria volontà con decisione giurisdizionale definitiva, ribadita dalla sentenza n. 334 del 2008 della Corte costituzionale in riferimento ad un temerario conflitto di attribuzione sollevato da Camera e Senato. Avremmo, quindi, la paradossale situazione in cui l'ordinamento riconosce un diritto ma esso non può essere esercitato, ciò pare in contrasto con i principi generali dell'ordinamento stesso; la negazione di ogni stato interpretativo aperto, affidato al medico e avuto riguardo alla volontà del paziente (ovvero del fiduciario che lo rappresenta), la non assimilazione *a priori* ed in forza di legge dell'idratazione e dell'alimentazione al trattamento o all'accanimento terapeutico, l'equiparazione della particolarissima situazione dello stato vegetativo permanente a tutte le le situazioni cosiddette "di fine vita", non certo assimilabili le une alle altre, il diretto e voluto contrasto con la sentenza n. 21748 del 2008 della Cassazione e con i pareri del Comitato Nazionale per la Bioetica (resi, in materia, nel 2003, nel 2005 e nel 2008) il mancato riguardo alle condizioni soggettive di ciascuna persona coinvolta, l'indeterminatezza dei termini e dei soggetti obbligati, rendono la norma irragionevole, sproporzionata ed abnorme, nonché configgente con l'articolo 32 della Costituzione e con i principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (si veda da ultimo la sentenza n. 438 del 2008 e, ancor prima, la sentenza n. 238 del 1996),

in esame riproduce i contenuti di un provvedimento di decretazione d'urgenza per il quale è stata valutata l'insussistenza dei requisiti per l'emanazione ai sensi dell'articolo 87 della Costituzione. I profili di illegittimità costituzionale che i senatori del Partito Democratico, in modo unanime, hanno rappresentato in sede di esame per il parere nella Commissione affari costituzionali riguardano due ordini di ragioni. La prima ragione è che noi riteniamo che il disegno di legge sia privo del requisito, e sia e sia anzi in manifesto contrasto, con il principio di ragionevolezza in quanto, il disegno di legge detta una disciplina a carattere esplicitamente provvisorio nello stesso identico momento essa è temporalmente indeterminata: quindi, una disciplina provvisoria a tempo indeterminato. Questa previsione non solo fa a pugni con la logica ma rischia, ciò che è ancora più grave, che la completa e organica disciplina legislativa in materia di fine della vita, in una materia così sensibile qual è la tutela dei diritti della persona, entri in contrasto con il combinato disposto degli articoli 3, 13, primo comma, e 32, secondo Tanto è vero, signor Presidente, che si dice che sia stato presentato un emendamento, anche se a firma di colleghi parlamentari, che pone già un termine al provvedimento. Ma il testo di cui noi iniziamo l'esame in questo momento è un testo, ovviamente, che prevede che la disciplina provvisoria sia a tempo indeterminato. Colleghi, il profilo assai più grave - lo voglio ricordare -che il Presidente della Repubblica ha inteso sottoporre alla valutazione del Presidente del Consiglio dei ministri) riguarda il fondamentale principio della distinzione e del reciproco rispetto tra poteri e organi dello Stato. È un principio che non è soltanto alla base della Costituzione repubblicana: il principio della separazione dei poteri è uno dei principi fondamentali di qualunque Costituzione democratica. Il Governo ha osservato, nel disegno di legge e nella relazione che lo accompagna, che vi è un profilo di questo tipo e ha inteso sostenere che la decisione della Corte di cassazione, in quanto disposta nella forma non di una sentenza,

Al contrario, colleghi, sappiamo perfettamente che la Suprema Corte ha più volte affermato che le decisioni della Corte di cassazione hanno ad oggetto diritti soggettivi costituzionali e non ammettono ulteriore impugnabilità nel merito. Per queste ragioni, evidentemente, la motivazione con la quale il Governo nella relazione di accompagnamento pone il problema e ritiene di superarlo appare assolutamente incongrua. Per queste ragioni, signor Presidente, oggi oggi siamo di fronte certamente ad uno dei momenti più delicati della vita di questa legislatura. Siamo convinti profondamente, senza entrare nel merito e prima ancora di entrare nel merito, che vi sia qui un tentativo ed un *vulnus* gravissimo non solo alla lettera ma anche allo spirito della Costituzione. Per queste ragioni, signor Presidente, i senatori del Partito Democratico chiedono ai colleghi e all'Aula di deliberare, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1369.

senza entrare, in questa fase, nel merito dell'esame del provvedimento, perché questa è una fase nella quale alcuni colleghi hanno sollevato una serie di questioni di costituzionalità del provvedimento che dal nostro La prima questione sollevata riguarda la circostanza che il contenuto del disegno di legge di iniziativa del Governo riproduca esattamente il contenuto del decreto-legge rispetto al quale il Capo dello Stato ha interposto un diniego all'autorizzazione e alla pubblicazione. credo che proprio questo dovrebbe farci riflettere, perché il rapporto fra il Governo e il Parlamento e il rapporto fra il Governo e il Capo dello Stato, soprattutto nella fase eccezionale dell'esercizio del potere normativo da parte dell'esecutivo, è un rapporto che la Costituzione disciplina in una maniera chiara e che non ha bisogno di essere né interpretato né forzato strumentalmente. Questo riguarda

e non entro nel merito, perché ogni decisione, per carità, è criticabile, che non vi fossero i presupposti di cui all'articolo 77 per procedere con decretazione d'urgenza e ha indicato la strada alternativa. Il Governo aveva due possibilità, o sollevare il conflitto dinanzi alla Corte costituzionale o proporre al Parlamento di esaminare la questione. Ritengo che la seconda sia costituzionalmente la più corretta, considerato che il Parlamento già si sta occupando della questione e che, proprio perché si tratta di diritti fondamentali che attengono alla dignità della persona umana e alle sue libertà fondamentali,

corretto e coperto integralmente dalla Costituzione. E grazie a Dio che ce l'abbiamo questa Costituzione, che non è il caso di cambiare soprattutto su questi aspetti, perché consente di ricondurre nell'ambito

perché casi simili a quello della povera Eluana oggi in Italia sono stimati nell'ordine di un paio di migliaia. È chiaro che ogni caso ha una storia clinica a sé. Nessuno vuole equiparare, non ho la competenza né la professionalità

sulla questione se nell'ambito del trattamento medico debbano essere ricomprese, quindi suscettibili di valutazione discrezionale ai fini della sospensione,

Al di là del rispetto umano che si deve alla famiglia e della circostanza che non sia giusto esprimere giudizi, che attengono a scelte e a situazioni che in ciascuna famiglia possono

dalla pregiudiziale di costituzionalità che è stata presentata, che non si può far diventare un provvedimento di volontaria giurisdizione, solo perché apprezzato dalla Cassazione, un provvedimento con gli stessi caratteri della sentenza passata in giudicato.

non hanno contraddittorio pieno e, sotto il profilo dell'accertamento e della cognizione del fatto, recano all'interno una valutazione parziale. Il che li rende, per loro

che hanno la responsabilità di natura sanitaria sotto il profilo dell'assistenza dovevano attenersi. La prima questione riguarda l'irreversibilità dello stato del paziente, e la circostanza che si faccia riferimento all'irreversibilità significa che non si può andare attraverso un giudizio che guardi all'alta improbabilità della cosiddetta reversibilità: poiché lo stato di salute del paziente deve essere tale da poter essere ritenuto irreversibile con esclusione di qualsiasi margine di dubbio, questo è il primo metro a cui il giudice della volontaria giurisdizione si deve attenere. Il secondo è l'accertamento

non sta a me dirlo sotto il profilo tecnico, scientifico e medico - possono essere rimessi in discussione. Da qui la natura del provvedimento stesso. Rispetto a questi casi, poiché l'articolo 32 della Costituzione recita che "Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge", "per disposizione di legge" significa, dal nostro punto di vista, che non può essere né un magistrato, né un terzo (sia il padre o sia un parente) a decidere per la persona malata. È la legge che decide e il Parlamento che lo fa stabilendo regole e criteri, che siano equi, giusti e conformi ai princìpi di tutela della dignità della persona umana; ma è sempre il Parlamento che interviene con legge, caro collega Bianco. Allora aggiungo, caro collega Bianco, che voi non avete il coraggio di dichiarare quello che pensate su questo provvedimento e vi trincerate dietro questioni regolamentari, procedurali e di presunta incostituzionalità senza dire se per voi

Presidente, il tema che avevamo sollevato all'inizio, ossia che non era stato distribuito il testo delle questioni pregiudiziali, è quanto mai importante visto che il senatore D'Alia evidentemente non ha letto le nostre pregiudiziali di costituzionalità in cui chiariamo che l'idratazione e l'alimentazione sono trattamenti medici sanitari che si possono e si debbono poter rifiutare. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo della Lega Nord esprimerà un voto contrario sulle questioni pregiudiziali proposte. Al di là della complessità del caso che stiamo valutando e del provvedimento che andremo ad adottare,

In sintesi, promuovono una lettura della Carta costituzionale diretta a riconoscere una sorta di diritto alla non cura, che significa in fondo il diritto di morire. Noi crediamo invece che la nostra Carta costituzionale non promuova il diritto di morire, che la morte non sia una manifestazione del diritto alla salute, ma che sia esattamente il contrario. La salute dell'individuo, oltre che un bene personale dell'individuo, è un interesse della collettività e la nostra Costituzione non ammette assolutamente che si possa

la nutrizione e l'idratazione non sono trattamenti medici, non sono accanimento terapeutico, ma sono atti dovuti eticamente e deontologicamente. Ci sono dei medici che - com'è successo pochi giorni fa - hanno fatto una serie di levate

Il mio Gruppo voterà contro le questioni pregiudiziali e si accinge a pronunciare due sì: sì ad una legge che ribadisca il principio fondamentale di indisponibilità della vita umana, sempre e comunque degna del massimo rispetto e del massimo sostegno; sì ad a una legge per Eluana,

Signor Presidente, oggi in quest'Aula si chiude un cerchio che in questa stessa Aula si è aperto dopo quella che è stata impropriamente chiamata la sentenza della Corte di cassazione. Ha ragione il collega D'Alia quando afferma che trattasi di un procedimento di volontaria giurisdizione. Tutti noi ricorderemo che siamo stati chiamati, prima della pausa estiva, a discutere di un possibile conflitto di attribuzione e che la nostra proposta è stata giudicata irricevibile dalla Corte costituzionale. Noi notavamo che in quella sentenza, in quel procedimento di volontaria giurisdizione, fossero almeno tre princìpi che fuoriuscivano dal nostro ordinamento e che per questo motivo quell'atto non giungeva soltanto a coprire un vuoto normativo, ma faceva molto di più. Innanzitutto, fissava la possibilità di ricostruire la volontà su base indiziaria, riferendosi a dichiarazioni e addirittura a stili di vita. Stabiliva inoltre che idratazione e alimentazione debbano considerarsi cure, contravvenendo in questo modo non solamente a quella che è un'acquisizione della maggioranza della scienza medica, ma anche a un dato di civiltà, in rispetto del quale in Occidente acqua e cibo non si negano nemmeno alle piante o ad altri esseri vegetali. Infine, invertiva l'onere della prova, affermando che il medico può intervenire solo in caso di consenso informato. Dunque, sulla base dei due princìpi precedenti, se non c'è o non si ricostruisce un atto che consente idratazione e alimentazione, il medico ha le mani legate. Signor Presidente, vorrei far notare anche ai colleghi

tema del fine vita, neanche quelli più distanti dai convincimenti di chi parla, avrebbe consentito ciò che sta accadendo a Udine.

mi chiedo e chiedo ai colleghi dell'opposizione: veramente si pensa che il Parlamento possa rimanere estraneo? Veramente si pensa che, di fronte ad un atto che ha una siffatta profondità culturale e giuridica, i rappresentanti del popolo - quali noi siamo - possano astenersi dall'assumersi le loro responsabilità?

Ci è stato detto di no, ma non nel merito, solamente per una questione di forma, quando abbiamo chiesto un conflitto di attribuzione alla Corte costituzionale. sempre senza entrare nel merito, quando ha messo in discussione alcune parti di quell'atto di volontaria giurisdizione. Infine, è stato detto di no quando il Governo si è preso la responsabilità di emanare un decreto. Questa è la verità ed è per questo che non vorremmo sentire più in quest'Aula il *non possumus*. Si è detto che in questa fase della discussione non dobbiamo entrare nel merito, nel merito, ma il merito di questa vicenda e di quello di cui parleremo nelle prossime ore, signor Presidente, è che cosa considera ognuno di noi per vita e che cosa considera ognuno di noi per libertà.

non solo sbagliato, ma anche vigliacco coprirsi dietro la Costituzione. Si discuta nel merito, ognuno si assuma le proprie responsabilità e si prendano determinazioni su un atto che segnerà la vita del nostro Paese per decenni.

non metto in votazione nulla se non siete tutti seduti. Metto

nella libertà di ciascuno di scegliere secondo i propri valori, secondo la propria coscienza e, eventualmente, secondo la propria fede a quali condizioni vivere e a quali condizioni morire. Pochi anni fa, una persona è morta tra le mie braccia dopo mesi di sofferenze indicibili che le hanno tolto progressivamente la mobilità, l'autonomia delle funzioni, la parola, il sorriso e, infine, il respiro e che, prima ancora della vita, le hanno tolto, giorno dopo giorno, la dignità della vita. Penso a quel poeta che diceva "Evitiamo la morte a piccole dosi ricordando sempre che essere vivo richiede uno sforzo molto maggiore del semplice fatto di respirare".

ma oggi non si discute di questo. Si discute di una norma ponte verso la possibilità di una legge, una norma che proprio per la complessità e delicatezza della materia, considerato che siamo ormai vicini ad una sua organica disciplina giuridica, ci suggerisce, in attesa di essa, di astenerci da atti irreversibili su cui si dovrebbe sospendere il giudizio, atti che, certo con il nobile intento di lenire il dolore ma anche con il discutibile arbitrio di saperlo interpretare correttamente, gettano ponti assai fragili e instabili sul vuoto della legge. Così va letto il pur lodevole tentativo di una sentenza di una corte di giustizia che, al di là delle buone intenzioni, di fatto introduce la possibilità per il nostro sistema sanitario

la politica rispettasse il dolore e se ne tenesse più lontana.Oggi la politica, per dirla con Pessoa, è un calice che trabocca di dolore altrui e ciò non avrebbe dovuto essere. Per questo motivo il buonsenso, l'incertezza, la discrezione, l'umiltà di fronte alla morte mi spingono ad esprimere un voto favorevole, che sento come un male ma comunque un male minore rispetto al grande male di questoperdurante, insopportabile vuoto nel quale compaiono inquietanti mostri.

Grazie, Signor Presidente, uso il poco tempo disponibile per motivare il mio voto contrario. Una decisione difficile, certo, forse la più difficile che ho dovuto prendere da quando sono in Parlamento, ma in coscienza non mi sento non mi sento di fare diversamente. La maggioranza ha voluto sottrarre al Parlamento il diritto di discutere nel merito su questioni di grande complessità, sul difficile incrocio di diritti individuali e di valori collettivi, sulla capacità di ricavare un unico diritto dal pluralismo etico proprio di un Paese. Ci viene chiesto semplicemente di arruolarci in una sorta di guerra civile. Rifiuto questo arruolamento. II Paese avrebbe invece bisogno di una classe politica capace di costruire le ragioni di una pace civile, a maggior ragione in materie che toccano così da vicino le coscienze individuali. Ci sarebbe bisogno, in queste materie, di leggi che vengano sentite tali da tutti i cittadini, non di manifesti ideologici. Le ultime scelte del Governo vanno oltre le scelte di merito. Si sta esercitando attorno al povero corpo di una donna un macabro esercizio senza pietà e senza rispetto della dignità umana. Un corpo, una persona che meriterebbe rispetto diventa l'oggetto di un puro gioco di potere. Chi crede che nell'azione del Governo sia in gioco la difesa della dignità della vita umana non può non vedere che quello stesso Governo, poche ore prima, ha fatto approvare una norma che, ad esempio, impedirà ad una donna che già vive il peso della clandestinità

Non c'è niente di peggio quando l'animosità dei convertiti si unisce al cinismo di un potere insofferente delle regole. Ho visto il Governo mandare degli ispettori alla ricerca del cavillo giuridico; questo in un Paese dove si muore, signor Ministro, per malasanità, dove in tante parti del Paese non c'è il diritto alla sanità e non vengono mandati gli ispettori. Avete avuto tanti mesi per arrivare ad una soluzione ragionevole, possibile con una legge che avrebbe potuto avere un ampio consenso. Per vostra responsabilità questa legge non è stata fatta ed ora fate un provvedimento che aprirà probabilmente altri dolorosi contenziosi. Trovo offensive e vergognose le parole del Presidente del Consiglio: "Eluana potrebbe avere un bambino", ed altri particolari che mi vergognerei a ripetere. Non avete rispetto per la persona, per la donna, per la famiglia, per le migliaia di famiglie italiane che accudiscono i propri cari in stato vegetativo, spesso senza alcun aiuto da parte dello Stato. *(Applausi dal Gruppo con le sofferenze di familiari malati terminali, di dolorose decisioni molto concrete sul confine della vita e della morte in cui le certezze dei teologi e l'opportunismo dei politici sono di poco aiuto. Sono grato al Presidente della Repubblica perché ha difeso senza incertezze la nostra Costituzione. Anche questo è un valore importante. La democrazia non è un orpello retorico, ma è lo strumento necessario per la costruzione del bene comune. Il valore così grande della vita non è mai stato garantito nei regimi totalitari. Termino per dire che non esprimo voto favorevole anche per una forma di civile protesta contro quella mancanza di umanità che ha caratterizzato troppi protagonisti di questa vicenda, quella virtù che sul piano civile si chiama pietà, che per i cristiani dovrebbe diventare carità. Sono virtù che fanno grandi una Nazione. Quando la politica e la religione pensano di farne a meno chi ne soffre è tutta la comunità nazionale.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, negli occhi di coloro che si sono espressi a favore di questo provvedimento, si scorge la pericolosa strumentalizzazione di una triste vicenda umana. La Costituzione italiana non risolve tutto, ma sancisce princìpi inderogabili: la libertà dell'individuo, l'inviolabilità dei suoi diritti nonché la separazione dei poteri dello Stato. Ma la volontà dei sostenitori di questo provvedimento non è quella di affrontare e risolvere una problematica di rilevante interesse sociale bensì quella di contestare e contrastare le decisioni del potere giudiziario creando un pericolosissimo ed inaccettabile precedente. Un attentato al fondamentale e democratico principio della separazione dei poteri attuato al solo fine di consacrare l'onnipotenza del Governo e dei suoi membri. Nessuna sentenza potrà più dirsi certa ed irrevocabile, perché il Presidente del Consiglio potrà decidere il contrario con il provvedimento che riterrà più comodo e per sé più utile. Si è attuata un'aggressione senza precedenti, anche nei riguardi del Presidente della Repubblica e delle sue funzioni, qualificate dal *Premier* come formalismi, disconoscendone il ruolo di guida e l'importante compito di garante dei requisiti di costituzionalità di ogni provvedimento. Non si possono ignorare a cuor leggero le obiezioni del Capo dello Stato, ma anche questo non interessa a chi si crede onnipotente. Questo provvedimento *ad personam*, dunque, è uno strumento vile, concepito in modo subdolo e sleale, strumentalizzando e sfruttando senza vergogna il caso drammatico di Eluana e della sua famiglia, in sfregio alla Costituzione, al Presidente della Repubblica ed al potere giudiziario. Approfondendo il merito della questione, è lampante, ancora una volta, la volontaria violazione della nostra Carta costituzionale. Non è poi vero che in caso di incapacità del malato di manifestare la propria volontà non siano presenti indici normativi di riferimento per giungere alla risoluzione del problema. L'articolo 9 della Convenzione di Oviedo chiarisce che è necessario, quando il soggetto non è più in grado di esprimere la propria volontà, tenere in considerazione i desideri dallo stesso precedentemente espressi. Certo, non è pensabile che chi non rispetta la Costituzione, non rispetta il potere giudiziario, non rispetta il Capo dello Stato, non rispetta il dolore altrui, rispetti invece una Convenzione ratificata nel lontano 1997. Come cattolico mi rammarico allora nel dover censurare posizioni proprie anche delle istituzioni religiose, ma ricordo come Papa Giovanni Paolo II, giunto al confine della vita, rifiutò l'accanimento terapeutico, chiedendo con umiltà di essere lasciato tornare alla casa del Padre. Per tali ragioni, ritenendo vergognoso che tale questione sia approdata in Parlamento in questo modo, esprimo il mio voto contrario.

quest'Assemblea, l'opposizione discute di altro. Qui al Senato ci sono due Gruppi, tra loro contrapposti, rispetto al tema oggetto di questo disegno di legge, ma finora abbiamo sentito dal Partito Democratico e dall'Italia dei Valori disquisire rispetto all'opportunità costituzionale di un intervento, criticare la politica sanitaria e

Mi ha stupito che, da una parte, si

alla volontà di portare a compimento un provvedimento e, dall'altra, si annunci che il proprio Gruppo avrà libertà di voto secondo coscienza.

e contro una possibile valutazione e interpretazione terza di cosa sia la qualità della vita voteranno il nostro Gruppo e il nostro schieramento. contento di appartenere ad uno schieramento politico e ad un partito che oggi voteranno per la difesa della vita. E sono certo che, al di là delle quisquilie e al di là delle schermaglie e del voler sviare il dibattito dall'essenza del problema su cui oggi siamo chiamati (con una votazione peraltro dolorosa) a pronunciarci, questo consenso a favore della vita avrà una portata più alta e più ampia rispetto alla maggioranza che sostiene il Governo e che, legata a questo Governo, ne sostiene con convinzione anche il disegno di legge che oggi discutiamo. Signor Presidente, cari colleghi, in questi mesi, come è mia abitudine, ho molto ascoltato. Ma oggi mi sento moralmente in dovere di prendere la parola. Vi parlo per ciò che sono io, per quello che rappresento per i cittadini: un medico, un uomo di scienza che, per più di è stato vicino ai malati di cancro (che ha aiutato a guarire e a vivere a lungo, molto a lungo), ma vicino anche alla sofferenza, al dolore, alla morte. Per questo da molti anni ho lanciato il movimento per il testamento biologico e, su questo argomento, ho scritto quattro libri (non uno, ma quattro libri), per un totale di 2.000 pagine. Perché il tema è complesso, è difficile, è delicato. Per questo sono sconvolto oggi. Sono sconvolto dalla singolare, direi assurda, procedura cui stiamo assistendo. Una legge dello Stato, che riguarda la libertà individuale verrebbe sbrigativamente approvata sull'onda delle emozioni sollevate da un caso mediatico. Perché questo è il caso di Eluana: un caso mediatico, perché non ha nulla di diverso, dal punto di vista scientifico e umano, da altre centinaia di casi di coma vegetativo permanente nel nostro Paese, di cui nessuno si occupa. Dietro a una legge emanata per Eluana non ci sarebbe, dunque, né logica, né razionalità, ma essenzialmente un'onda emotiva, che per sua natura è passeggera e, soprattutto, è una cattiva consigliera.

per evitare di affrontare lucidamente il problema. Si tratta di un problema di civiltà, che riguarda l'invasione della tecnologia medica nella vita umana. Mi trovo d'accordo con il filosofo cattolico, cattolicissimo, Giovanni Reale, quando vede nel caso di Eluana ‑ sono sue parole ‑ un abuso da parte di una civiltà tecnologica che vuole sostituirsi alla natura. Quando avverte che si è perduta la saggezza della giusta misura e la Chiesa e il Governo sono vittime di questo paradigma dominante, che vorrebbe tenere in vita Eluana contro la natura e, infine, quando cita Papa Wojtyla, che, rispondendo ai medici che gli offrivano di continuare a curarlo, disse: «Lasciatemi tornare alla casa del Padre». un complesso di organi e cellule in una vita artificiale è un atto contro natura: tecnologicamente oggi la medicina è in grado di mantenere in stato vegetativo un corpo senza attività cerebrali quasi all'infinito, ma il fatto che lo si possa fare tecnicamente non significa che lo si debba fare eticamente. Penso sia una mostruosità, e come me la pensano migliaia e migliaia di cittadini, terrorizzati dalla prevaricazione violenta della medicina tecnologica nella propria vita. Lo dico da uomo di scienza: la tecnologia non ha limiti in sé, e se noi, la società e le sue istituzioni non ci impegniamo a tracciare questi limiti rispetto alla vita dell'uomo, chi mai lo potrà fare? Conosco bene la normativa italiana sul diritto di cura, perché ogni giorno la applico e la vivo insieme ai miei medici e ai miei malati: la nostra legge garantisce la possibilità di rifiutare ogni trattamento, anche di semplice sostegno, come le trasfusioni di sangue e la nutrizione artificiale; abolire questo diritto sarebbe un atto molto grave, che minaccia alle radici il principio di libertà individuale, base irrinunciabile delle democrazie moderne. Voglio pertanto fare un appello alla ragione e alla coscienza di tutti noi e di tutti voi, in quanto membri del Senato, vale a dire di questa Camera alta, di questa istituzione a cui la gente guarda come un punto fermo nella confusione dei momenti di crisi: il nostro ruolo è di analizzare le situazioni più difficili con lucidità e saggezza e dare pareri obiettivi e lungimiranti. Ecco, credo sia nostro dovere, come senatori, guardare più in là dell'oggi e anche del domani e pensare anche alle conseguenze future delle nostre decisioni. Vi chiedo, dunque, di fermarvi, di riflettere, di meditare e di non votare una legge in palese contrasto

di poter rifiutare quella condizione assurda ed inumana di una vita artificiale, che può protrarsi per decenni, priva di coscienza e di attività cerebrale. Bene, al contrario, questo provvedimento imporrebbe a tutti, per legge, proprio questa fine terribile e innaturale. *(Vivi,

Signor Presidente, signori membri del Governo, colleghi senatori, la vicenda drammatica di Eluana Englaro ha colpito molto il Friuli-Venezia Giulia, una Regione tranquilla, ferma nei principi collettivi, nei valori cristiani e nelle tradizioni condivise che hanno saputo unire le persone nei momenti più difficili. Come nel 1976, quando nel terremoto morirono migliaia di persone, mettendo in ginocchio l'intero sistema sociale, e la Regione si trovò a dover far fronte ad un dramma comune e al mistero di una morte collettiva, che aveva portato via intere famiglie, bambini, mamme, papà, anziani. Da quella data sono passati trentatré anni e oggi il Friuli, forte di quelle tradizioni antiche, ma sempre attuali, si trova in primo piano nella triste storia di Eluana Englaro. La nostra società sta attraversando un momento di crisi dei valori in cui la precarietà e la vulnerabilità prevalgono sulla stabilità e le certezze delle persone che, alla profondità della riflessione, preferiscono troppo spesso la superficialità, figlia delle scelte immediate, ma non ragionate. Pertanto, il dibattito sulla commovente vicenda Englaro non può essere «questione privata», come è stata definita da alcuni. La vita e la morte hanno sempre una natura collettiva; possono essere privati i sentimenti che l'accompagnano (e non entro nel merito del dolore di un padre e di una madre che si trovano di fronte a una scelta così difficile), ma non sono privati i principi che uniscono le persone e le comunità. La vita, intesa in ogni sua forma, non è una cosa privata per definizione (anche se sul caso vi è stata un'attività eccessiva da parte dei *media)*, così come non è esclusivamente privata la ricerca del senso nei percorsi di ognuno di noi verso gli altri, in cui la missione che ci viene affidata ha un significato collettivo e non soltanto individuale. La vita di Eluana Englaro ha un senso collettivo che sta coinvolgendo milioni di persone che in quella scelta, nel rispetto del dolore dei familiari, ricercano significati e speranze anche per ritrovare quella missione che, da cristiano e cattolico, ritengo Dio abbia assegnato ad ognuno di noi. In questo momento, anche se triste, l'auspicio è che ritornino talune centralità sul diritto alla vita, che va rispettata in ogni sua forma e accettata e compresa anche quando tutto questo diventa difficile da vivere e da comprendere. Ringrazio il Governo per l'iniziativa assunta, in particolare il ministro Sacconi per l'impegno che ha profuso insieme al Sottosegretario nelle ultime settimane, e manifesto il mio consenso alla proposta del Governo.

Presidente, onorevoli colleghi, il tono e la qualità del dibattito in alcuni interventi mi auguro abbiano suscitato in tutti i presenti, come in me, in chi vi parla, motivi di riflessione e di approfondimento su una tematica - lo hanno detto in tanti, lo avvertiamo tutti che definire complessa è riduttivo. Ho apprezzato molto l'intensità dell'intervento del professor Veronesi, come di Paolo Giaretta, e li ho apprezzati ancora di più perché dopo l'intervento sono rimasti in Aula ad ascoltare, a testimonianza - ahimè, siamo in pochi che la profondità di queste tematiche necessita innanzitutto di una capacità di confronto e di ascolto che purtroppo qualche volta manca. Voglio ricordare a me stesso e a tutti noi che nel mese di luglio quest'Aula approvò all'unanimità un ordine del giorno in cui ci impegnammo, l'Aula del Senato si impegnò, a legiferare sulle disposizioni anticipate di trattamento entro la fine dell'anno. Se vi avessimo ottemperato, oggi vivremmo qualche angoscia in meno; non mi sento di poter dire qualche certezza in più, ma comunque saremmo più tranquilli perché in qualche modo avremmo ottemperato a quell'impegno che avevamo assunto in quest'Aula. C'è un contesto che appesantisce questa vicenda che io cerco di non limitare o perimetrare come il caso di Eluana Englaro, perché riguarda Eluana Englaro, ma non solo. Lo ricordava bene il professor Veronesi: ci sono migliaia di di esseri umani che vivono questa condizione. Quindi io vorrei, dopo qualche premessa, entrare nel merito del provvedimento, del testo con il quale ci confrontiamo, delle domande essenziali, sostanziali alle quali ciascuno di noi deve rispondere in piena coscienza. Io respingo il bipolarismo dei valori o il bipartitismo delle coscienze che anche qui appesantisce e sconfigge, su queste tematiche, la politica. Essere esponenti della maggioranza o dell'opposizione, come chi vi parla, non deve incidere, sostanzialmente, rispetto a questa discussione e alle tematiche eticamente sensibili, quelle rispetto alle quali ciascuno di noi si forma un'opinione nel convincimento e nel confronto tra laici credenti e non credenti, consapevoli come dobbiamo essere che non esiste il monopolio rispetto a questi valori, né di una categoria né dall'altra. Certamente, quello che sta accadendo in queste ore ma anche nei mesi precedenti, lo scontro che caratterizza l'approccio a questo dramma umano e familiare non ci aiuta a riflettere. Diciamo comunque, senza ipocrisie e conformismi, che la spettacolarizzazione di questa vicenda muove anche - lo dico con rispetto vero e autentico

ha elevato questo dramma e lo ha portato in altri terreni e in altri territori. Allora, tutti parliamo di silenzio, di cautela, di prudenza, però alla fine i primi che propongono silenzio, cautela e prudenza poi disattendono queste premesse che invece sarebbero indispensabili principalmente per favorire ed esaltare la capacità di ascolto nel confronto.

precisando in premessa il pieno rispetto di tutte le posizioni che con grande onestà intellettuale e con grande intensità sono state rappresentate fino adesso in quest'Aula, che sono quelle che leggiamo quotidianamente e ascoltiamo. Come spesso accade, su queste tematiche ognuno di noi si forma un'opinione ascoltando, leggendo,

siamo quasi in contraddizione con noi stessi perché il tema è oggettivamente difficile e non lo si può affrontare né in punto di diritto, né in punto di procedura e - ahimè - nemmeno in punto di scienza. È un mistero il caso che viene compreso in questo disegno di legge che, ripeto, non si esaurisce in questo. Una ragazza che da diciassette anni vive questa condizione e che non sviluppa stati infettivi, non presenta piaghe da decubito, leggo che ha ancora i ritmi di sonno e veglia e altre funzioni vitali: questo è un mistero, se si vuole, dovuto sicuramente anche alle amorevoli cure di chi assiste da diciassette questa povera sventurata, però è anche un qualcosa che scientificamente deve farci interrogare. Quella condizione, quella posizione, tutto questo è terreno - ahimè - fertile per portarla via per altri motivi. Non c'è un respiratore meccanico che funziona, non c'è la morte cerebrale, altrimenti forse avrebbero provveduto all'espianto

ma l'idratazione e l'alimentazione parentelare in un organismo che per vivere non ha bisogno di respirazione artificiale e di ausilio è accanimento terapeutico

siano molte le condizioni in cui un essere umano non sia in condizione di assumere liquidi e di alimentarsi. il mio approccio da tutto quanto lo appesantisce e rappresenta una sconfitta della politica, perché noi avremmo dovuto licenziare una legge che al proprio interno

affermativamente è se l'alimentazione parentelare (il sondino, l'idratazione) sia un sostegno vitale. Io rispondo sì, per me è un sostegno vitale. Non vorrei, con questa affermazione, essere in qualche modo in qualche modo catalogato tra quelli che si mettono da una parte e in contrapposizione all'altra. adesso una notizia triste, rispetto alla quale non posso far altro che interrompere il mio intervento. Non lo concludo perché le nostre considerazioni sono purtroppo superate dalla tragica attualità.

Colleghi, non mi pare sia questo il modo per

desidero esprimere la partecipazione di tutti i membri del Governo al grande dolore dei familiari di Eluana Englaro di tutte le persone che le sono state vicine, in particolare in questi lunghi diciassette anni. Abbiamo sempre comprensione per le scelte del padre di Eluana Englaro, anche se non ne abbiamo condiviso lo scopo. In questo momento ricordiamo anche quelle suore misericordine che si sono, a lungo e con straordinario amore, prese cura di lei, persona viva fino a poco fa ed ora deceduta. Nell'esprimere, come ho detto, la partecipazione di tutti i componenti del Governo, ma anche

affinché questo sacrificio non sia stato inutile del tutto e possa indicarci la strada, sia di un provvedimento tempestivo tempestivo sia di una disciplina più organica e compiuta alla quale questo stesso provvedimento vuole fare riferimento. Grazie, un laicissimo principio del dubbio che riguarda i tanti profili, soprattutto sostanziali, prima che formali, in nome del quale io mi auguro l'Aula vorrà considerare quel principio di precauzione in favore della vita che ha ispirato l'iniziativa del Governo per un decreto-legge, prima, e per un disegno di legge, poi.

dell'idea che il miglior modo per ricordare una persona che non c'è più sia quello di dare al Paese l'immagine di un Parlamento che comunque si assume delle responsabilità, non più sotto l'incalzare di una vicenda che ormai ha raggiunto un terribile epilogo, ma

A me spiace che l'iniziativa legislativa su questo delicato tema possa essere compiuta e realizzata in un momento così triste e doloroso. La nostra solidarietà e la nostra vicinanza al papà di Eluana le abbiamo sempre manifestate in tutti i nostri interventi. È un momento di grande dolore, è un momento in cui tutti noi siamo chiamati a riflettere. Tutti noi, componenti di un Parlamento che è chiamato ad assumersi le responsabilità sull'individuazione del confine del diritto alla vita e del diritto alla morte, abbiamo il dovere di essere non soltanto partecipi a questo doloroso momento, ma anche di decidere una volta per sempre. Facciamo in modo che il Parlamento, che è la casa degli italiani, possa continuare questo percorso per dare un segnale al Paese. Un Paese che ha bisogno di vedere nelle istituzioni un punto di riferimento; istituzioni all'interno delle quali si discute, si dibatte, ci si confronta, a volte ci si allontana, ma non dimenticando mai di tenere alto il principio del rispetto degli alti valori

Presidente, la ringrazio per aver riportato l'Aula a compostezza costo di non essere politicamente corretto, non voglio che passi che è successo un incidente. Noi dobbiamo considerare che dietro le scelte politiche ci sono delle persone umane, ci sono il sangue, i nervi, le speranze di persone in carne ed ossa. In questi giorni tutti hanno assunto delle decisioni politiche

la parola in un altro modo. Credevo di poter dire, a nome di tutti quelli che sono qui e che in qualche modo, con idee diverse, hanno partecipato alla discussione in quest'Aula, nella Conferenza dei Capigruppo e sui giornali, che questo è il momento in cui, come padri e come madri, visto che ci eravamo assunti questa responsabilità, piangiamo Eluana. Non è così. Viene compiuto, sulla morte di Eluana, l'ennesimo atto di sciacallaggio politico. *(Vivi Ministro Sacconi, ho apprezzato le sue parole, ma non posso apprezzare quelle del senatore Quagliariello. La straordinaria, bieca e volgare strumentalità con la quale il centrodestra e il presidente Berlusconi in prima persona hanno affrontato la questione ricade nel momento più triste.

Il tentativo che è nelle parole del senatore Quagliariello, quindi, si rivolge ad un profilo che è così alto e così grave nella nostra Repubblica da non poter essere tollerato.

La seduta è sospesa. convoco immediatamente la Conferenza dei Capigruppo.

Innanzitutto, ci si è confrontati sul significato delle espressioni del Vice Capogruppo di maggioranza, Grazie, su chi fossero i destinatari di quelle accuse ed il Vice Presidente del Gruppo, senatore Quagliariello, ha tenuto a ribadire come quelle affermazioni intendessero riferirsi ad un dato oggettivo

Per cortesia, quando avrò finito di parlare darò la parola ai Capigruppo. Sto riferendo all'Aula il contenuto di alcuni passaggi della Conferenza dei Capigruppo. È mio dovere e intendo farlo.

Vi sono state posizioni divergenti: vi è stata la posizione del Partito Democratico, che ha dichiarato di non voler più seguire il calendario e di volersi addirittura sottrarre all'esame di questo testo, ove si dovesse decidere di andare avanti;

vi è stata (e vi è) la proposta di mediazione della Presidenza, sulla quale non vi è stata convergenza, ma che ha delineato nuovamente uno scenario che vede la maggioranza e il Gruppo presieduto dal presidente D'Alia d'accordo

di affermare che il Parlamento, che aveva iniziato ad esaminare un testo di legge, non si ferma in relazione ad un fatto oggettivo, seppure drammatico e tragico, che colpisce tutti noi.

sull'esame dei testi di legge, così come era condiviso il percorso che stavamo attuando e realizzando, con l'assunzione di responsabilità da parte di tutti i Gruppi di maggioranza e opposizione.

per dire, con la pacatezza che è dovuta, che il Gruppo del Partito Democratico, che non condividerebbe la scelta di tornare a discutere di questo testo domani,

un articolato, in maniera tale da poter passare in tempi brevissimi alla discussione in Aula di un testo compiuto e - lasciatemi dire assai più soddisfacente sotto il profilo della previsione, della stesura, dell'approfondimento che lo ha accompagnato e che lo contraddistingue, in considerazione di un dato di fatto oggettivo. Stamattina il relatore di maggioranza in Commissione sul provvedimento che abbiamo in esame ha presentato un emendamento con il quale fissava in 180 giorni

dei problemi che la regolazione del fine vita solleva. Con la nostra proposta si recupera molto tempo rispetto a quei 180 giorni, con in più la possibilità di di giovarci di un lavoro già avanzato in Commissione e della disponibilità del mio Gruppo, che dei testi sul fine vita è stato autore, coautore e anche - lasciatemelo dire - portatore di ipotesi di mediazione rispetto a punti molto delicati. Credo che la nostra sia una proposta adeguata rispetto alla

di fissare perché il Parlamento adotti un atto di legislazione in questa materia. Davvero mi rivolgo

Anzi, torniamo a discutere sulla base non di un testo di parte, ma di un dibattito che si è dipanato solo in questa legislatura per sette mesi, che vede già un testo del senatore Calabrò e che ha raggiunto, con l'ulteriore sforzo che compiremo nelle prossime settimane, un punto di definizione che può soddisfare le forze di maggioranza e di opposizione.

vorrei dire ai colleghi che l'Italia dei Valori è contraria alla prosecuzione dell'esame di questo provvedimento che ha suggerito un ritorno immediato in Commissione perché si approvi in tempi definiti e stringenti il disegno di legge sul testamento biologico Lo dico per chiarezza, perché questa proposta nasce da un'esigenza che noi abbiamo inteso rispettare. Non abbiamo presentato alcun emendamento al disegno di legge del Governo e lo abbiamo fatto scientemente, proprio perché comprendevamo che il Parlamento dovesse assumersi la responsabilità in presenza di un caso, che è quello che aveva spinto - a nostro parere - il Governo e la maggioranza a indirizzarsi

e serio, manifestando il nostro cordoglio unanime nel momento in cui dobbiamo superare gli asti. Poi, ognuno di noi si assumerà le sue responsabilità e dichiarerà quanto dovrà dichiarare, ma in questa fase bisogna guardare all'obiettivo. Chi è credente rivolga una preghiera per una vita che non c'è più, chi non lo è faccia una riflessione. Credo, tuttavia, che dobbiamo avere insieme

Signor Presidente, c'è rabbia, tanta rabbia, perché questa morte si poteva sicuramente evitare. Un Paese civile Un Paese civile non può far morire una persona di fame e di sete. Questo è inaccettabile!

Signor Presidente, abbiamo apprezzato la sua proposta di mediazione e le riconfermiamo quello

della riflessione e, secondo noi, anche del rammarico per non essere arrivati in tempo a dare una risposta a questa vicenda. Però siamo anche consapevoli che vi sono altre 3.000

Quindi, noi riconfermiamo il nostro voto favorevole alla sua proposta di mediazione, che riteniamo l'unica possibile e che ci auguriamo venga accolta da tutti.

Ha chiesto di parlare il Governo nella persona del ministro Sacconi.

Presidente, colleghi, il Governo innanzi tutto conferma la propria convinzione circa l'urgenza con la quale deve essere garantita una regolazione, quantomeno nei suoi contenuti essenziali, della fine della vita, anche

l'opportunità di un percorso legislativo tale da garantire un esito in tempi certi di questa regolazione. La proposta che è pervenuta dal Gruppo del Partito Democratico, attraverso la sua Capogruppo, è è interessante nella misura in cui appare garantire il superamento di una situazione critica manifestatasi all'interno della Commissione, nella quale oltre 40 parlamentari si sono iscritti a parlare e altri potrebbero, in teoria, ancora prendere la parola.

che dovesse manifestarsi in termini ostruzionistici sull'intero provvedimento. Se la novità, come appare, è costituita dalla disponibilità dei Gruppi di opposizione a garantire un esame del provvedimento di regolazione della fine di vita, quale la Commissione sta esaminando sulla base di un testo base - chiedo l'ipotesi di avviare l'esame nelle prossime due settimane, con l'impegno, che mi sembra il Presidente del Senato voglia garantire come in altri casi ha saputo sempre garantire, di un *iter* certo dei lavori e, quindi, anche di modalità atte ad assicurarne non soltanto l'inizio ma anche il termine.

del quale il provvedimento presentato nei giorni scorsi e all'esame di quest'Aula costituisce, per il Governo stesso, un aspetto essenziale.

Signor Presidente, colleghi del Senato, membri del Governo, oggi abbiamo vissuto una giornata che certo non dimenticheremo facilmente ognuno di noi poi esprimerà opinioni e valutazioni. La norma che abbiamo oggi portato in quest'Aula era stata concepita, dal Governo che l'ha presentata, ma anche dal nostro Gruppo che era pronto a presentarne una analoga, come una norma ponte

Abbiamo preso atto di valutazioni altre. Chi ha assunto altre valutazioni lo ha fatto perché, evidentemente, riteneva di rispettare non solo la propria coscienza, ma anche la sua lettura della Costituzione repubblicana. I dibattiti di giuristi, costituzionalisti e di Presidenti emeriti hanno dimostrato, in questi giorni, che era lecito pensarla in un modo e in un altro e la letteratura è ampia al riguardo. Allora, siccome riteniamo che alcuni principi vadano scanditi... Sto parlando con grande rispetto, perché io sono una persona responsabile, cari colleghi del Senato! Una persona che difende la vita nel Senato della Repubblica, che è contro

È per questa ragione che propongo al Presidente di accettare la mia proposta di inserire all'ordine del giorno di domani mattina, lo dico anche agli altri Capigruppo, una mozione

che sancisca che l'idratazione e l'alimentazione non sono accanimento terapeutico e che non si può far morire nessuno di fame e di sete. *(Applausi dai Gruppi PdL e LNP)*. E questa mozione vogliamo che la voti il Senato domani, signor Presidente.

signor Presidente.

Signor Presidente, signor ministro Sacconi, prendiamo atto della proposta del Governo e della proposta,

Avremmo preferito, e continuiamo a preferire, un provvedimento avente forza di legge, che mettesse un punto su questa vicenda dobbiamo anche fare i conti con la logica dei numeri delle rappresentanze parlamentari, che rispettiamo. Pertanto, prendiamo atto che si è registrata una convergenza che almeno punta ad avere un clima più disteso nell'esame di questioni che meritano un maggior decoro, un maggior rispetto e anche una maggiore - mi si passi Detto questo, signor Presidente, se il collega Gasparri è d'accordo, intendiamo concorrere, come fatto con la proposta di legge, alla stesura di questa mozione, che ha un solo effetto (altrimenti non vorrei che cadessimo nell'equivoco), che di consentire al Parlamento, se non di fare una legge, di esprimere un pronunciamento politico chiaro, che sia un'anticipazione di ciò che fra due settimane ci auguriamo avvenga in quest'aula, ossia l'approvazione di un testo sulla legge di fine vita.

non si alza il livello dello scontro politico istituzionale a tal punto se poi non si è conseguenti con provvedimenti approvati dall'Assemblea, provvedimenti di legge. *(Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut e PdL).* Quindi, siamo qui e aspettiamo, prendendo atto delle sue dichiarazioni e di quelle del Presidente del Senato. Senato. Per il rispetto e la stima che abbiamo nei vostri confronti, siamo qui e condividiamo questo percorso, attenti affinché si possa realizzare anche con il nostro piccolo modesto contributo. Presidente, brevemente voglio esprimere il mio apprezzamento per lo sforzo che è stato fatto di superare un momento di grave tensione che, su una materia come questa, rischiava di creare un conflitto lacerante anche nella coscienza individuale e nel tessuto civile del Paese. Voglio esprimere, in modo particolare, il mio apprezzamento al ministro Sacconi... *(Applausi dai ha saputo essere capace, per quanto gelosamente appassionato della tesi che ha sostenuto e sulla quale ha determinato l'indirizzo del Governo, di una sensibilità istituzionale elevata, che è frutto anche della sua grande cultura politica. Conto molto su questo suo stile per giungere, nel concorso di tutte le forze parlamentari, ad una soluzione equilibrata di un tema complesso, nel quale chi rivendica certezze granitiche fa torto all'intelligenza e alla sensibilità degli altri. Presidente, trovo assolutamente ragionevole e la definirei appropriata la proposta che è stata fatta dal ministro Sacconi, che noi accettiamo. Mi pare legittimo che il Capogruppo del Partito della Libertà chieda di discutere domani mattina una mozione sui punti che riterranno essere quelli quelli desumibili dal testo che avevamo all'esame. Noi onoreremo il nostro impegno che abbiamo assunto in quest'Aula. Mi permetto di dire che credo di non dover ascrivere al merito, né mio né del mio Gruppo, ma dell'intera Aula di Palazzo Grazie, uno degli atti più sacri delle democrazie parlamentari, cioè una discussione vera, approfondita, seria, che ci conduca all'approvazioni in tempi brevi - come abbiamo promesso - di un testo sul fine vita.

e serena al problema che abbiamo davanti. Siamo convinti che insieme riusciremo a fare, pur nelle divisioni, pur nelle impostazioni differenti, una buona legge di cui il Paese ci ringrazierà.

Innanzitutto, chiudiamo questa drammatica giornata di oggi, lacerata dalla luttuosa e terribile notizia della morte di Eluana, con un impegno; un impegno di un Parlamento che dimostra, anche nei momenti più delicati, più conflittuali e più dolorosi, di riuscire con grande sforzo a trovare dei grandi momenti di sintesi. L'impegno che questa sera assume il Senato è quello di di definire e portare a termine un percorso del quale tante volte questa Presidenza ha parlato: quello di legiferare sulla normativa relativa al testamento biologico.